in data 9 ottobre 2006, è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri:* «Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania»

ricordare che ieri sera è venuto a mancare Nicola Matteucci, uno dei più grandi storici delle idee dell'Italia del secondo dopoguerra,

Il liberalismo di Matteucci ha attinto alla lezione anglosassone assai più che alla lezione continentale. Anche per questo è sempre stato nella sua vita un uomo di minoranza senza mai, però, essere un minoritario.

l'ha rappresentata in contesti nei quali questa era minoranza, come, ad esempio, all'interno della casa editrice «Il Mulino», che ha contribuito è stato uno dei collaboratori de «Il Giornale» di Montanelli, come tale anche corrispondente di altri filoni del pensiero liberale europeo, e penso ad esempio agli «anglofili» francesi di *Commentaire*, che l'hanno avuto attento interlocutore.

in adempimento, peraltro, ad una precisa prescrizione formulata nella risoluzione parlamentare di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria. Avevamo fatto bene allora ad impegnare il Governo alla presentazione - cito testualmente - «ove necessario, di una Nota di aggiornamento con le integrazioni al quadro degli elementi di ordine quantitativo concernenti in particolare l'entità e la composizione della manovra da realizzare per quanto concerne tanto gli interventi correttivi che quelli rivolti alla crescita ed all'equità sociale e territoriale». Il Governo ha adempiuto a tale prescrizione del Parlamento e oggi discutiamo una Nota di aggiornamento che affronta tutte le questioni indicate nella

Il primo si riferisce alle previsioni e all'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche. La Nota di aggiornamento registra il miglioramento dell'economia italiana nel corso del primo semestre di quest'anno. di una buona notizia che sappiamo dovuta al migliore andamento dei consumi interni ma anche, come ricordato dall'ISTAT, al recupero del settore estero. Nei primi cinque mesi dell'anno il fatturato industriale è aumentato del 7,2 per cento sul mercato interno e del 12,4 per cento su quello estero. Il miglioramento della congiuntura consente di correggere al rialzo la stima di crescita per l'anno in corso, che passa dall'1,5 per cento del DPEF all'1,6 per cento della Nota di aggiornamento. Ricordo che il DPEF aveva già registrato una previsione di miglioramento prevedendo l'1,5 per cento del PIL rispetto all'1,3 per cento della Relazione sull'andamento dell'economia del maggio 2006. Naturalmente si tratta di dati positivi, ma credo dobbiamo essere consapevoli che questi dati, su cui abbiamo in tanti fatto valutazioni anche positive, non ci possono dire che tutti i problemi sono risolti. Se la crescita rappresenta la sfida fondamentale dell'economia italiana, su cui negli anni passati abbiamo registrato pesanti *record* negativi - ricordo i due anni di crescita zero recenti dobbiamo essere consapevoli che i risultati positivi di questi primi mesi lasciano il problema del tutto aperto. Come ha ricordato il ministro Padoa-Schioppa, la crescita va misurata sui lustri, non sui trimestri. Il confronto europeo continua ad essere negativo per l'Italia, i nostri *partner* principali crescono più di noi ed è presto per dire quanto dell'attuale andamento ciclico positivo rappresenti un'inversione duratura rispetto all'andamento degli ultimi anni. La stessa Nota di aggiornamento ricorda che si prevede una moderazione nella crescita dell'economia nella seconda parte dell'anno. Quindi, i problemi di una politica economica capace di assicurare un'inversione di tendenza duratura sono tutti aperti e sono affidati alla capacità della legge finanziaria di incidere sul fronte dell'aumento della produttività totale dei fattori e della capacità competitiva del nostro sistema.

è giusto pensare a modifiche che ne migliorino gli aspetti negativi; tuttavia, l'impianto, basato su un'azione capace di restituire competitività al sistema delle imprese (la riduzione del cuneo fiscale, le azioni sul fronte dello sviluppo del Mezzogiorno, le azioni sul fronte dell'innovazione e della ricerca), rimane come dato positivo della strategia di politica economica del Governo. Il Il miglioramento congiunturale dell'economia italiana che ho ricordato e che la Nota di aggiornamento riporta è certamente all'origine del secondo dato che la stessa Nota di aggiornamento registra, e cioè l'evoluzione favorevole delle entrate. La Nota ci dice che ci troviamo in presenza di un miglioramento delle entrate erariali che, valutate in termini di anno, valgono circa 6 miliardi di euro rispetto a quanto previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria; tale aumento consente di rivedere in crescita le previsioni tendenziali delle entrate. Si tratta di un'inversione di tendenza netta rispetto agli andamenti degli ultimi anni, caratterizzati su questo fronte da una diminuzione che aveva assunto caratteri strutturali. E' un fatto positivo, si inverte un ciclo che era basato sulla diminuzione delle entrate e sull'aumento della spesa corrente, tuttavia non è certo il segno di un problema risolto. Le manovre della passata legislatura si affidavano in larga misura a provvedimenti di efficacia temporanea e il venir meno di queste entrate impone di tenere alta la guardia della manovra. manovra. Lo dico con riferimento alle discussioni di questi giorni sull'entità della manovra e richiamando il carattere strutturale della crisi dei nostri conti pubblici che il Ministro dell'economia ha ricordato illustrando la manovra alla Camera, evidenziando la forte espansione della spesa strutturale, che è aumentata di 2,6 punti di PIL nel periodo 2001-2005, l'aumento della spesa rigida, il Sistema sanitario nazionale, il pubblico impiego, i consumi intermedi, la scuola, il prosciugamento delle risorse per funzioni essenziali, come quella della realizzazione delle infrastrutture. Se è vero, quindi, come ci ricorda la Nota di aggiornamento, che ci troviamo in presenza di un miglioramento delle entrate, è altresì vero che in nulla incide tale aumento delle entrate sulle difficoltà strutturali dei nostri conti, dovute alle ragioni che ho ricordato. Il terzo punto su cui voglio brevemente soffermarmi è relativo ad una questione a cui la Nota di aggiornamento dedica una particolare attenzione. La Nota affronta il problema degli effetti sui conti pubblici della recente sentenza della Corte di giustizia europea sulla indetraibilità dell'IVA, aggiornando le previsioni tendenziali per l'anno in corso con riferimento a tale sentenza. Come è noto, la sentenza costituisce un riferimento molto importante e determina un significativo peggioramento delle maggiori grandezze di finanza pubblica. Ricordo che il DPEF prevedeva un indebitamento al 4 per cento e la Nota lo porta al 4,8 per cento, proprio per effetto della sentenza sull'IVA.

Ho ricordato ciò soltanto per sottolineare come la sentenza sull'IVA costituisca un ulteriore elemento di difficoltà a cui la manovra deve fare fronte. La sentenza era prevedibile dopo che la Commissione si era già pronunciata in modo chiaro sulla questione. Nella legislatura del centro-sinistra si erano avviate trattative per un graduale rientro nella regola europea e nel 2001, ricordo, era stata introdotta una prima correzione ai limiti di indetraibilità. Purtroppo, quel percorso di rientro è stato abbandonato nella scorsa legislatura. Oggi dobbiamo fare i conti con le pesanti ripercussioni sui conti pubblici, come ho ricordato citando le cifre. Il Governo ha affrontato questo problema; lo ha affrontato nell'apposito decreto-legge sull'IVA che dobbiamo convertire, lo ha affrontato nel decreto-legge collegato alla manovra, prevedendo la copertura delle maggiori spese derivanti da questa sentenza. Gli effetti di tali maggiori oneri sono stati registrati anche nell'aggiornamento del quadro tendenziale dei conti pubblici che il Governo ha presentato nel dibattito in Commissione, che ci consente oggi di avere un quadro piuttosto preciso di ciò che capiterà ai nostri conti.

La proiezione sul 2007 di 5 miliardi di maggiori entrate, aventi carattere strutturale, consente di ridurre l'entità della manovra necessaria per conseguire l'obiettivo di correzione dei conti indicato dal DPEF. L'effetto netto della manovra si riduce quindi da 1,3 punti di PIL ad un punto di PIL. Vengono confermati gli obiettivi del DPEF: indebitamento al 2,8 per cento, avanzo primario in progressivo aumento, fino a raggiungere il 4,8 per cento Il debito in rapporto al PIL è previsto in graduale riduzione, fino ad arrivare al 97,8 per cento nel 2011. La manovra, così come delineata, ha avuto un giudizio positivo in sede europea; riportano i quotidiani di oggi che il primo giudizio del responsabile della Commissione europea ha sottolineato come l'attuazione di questa manovra consenta ai conti pubblici italiani di andare strutturalmente sotto il 3 per cento, e quindi costituisca una risposta positiva alle esigenze di mantenimento degli impegni assunti in sede europea e del Patto di stabilità europeo.

ma il rispetto di tali impegni è un dato fondamentale; il risanamento dei conti nel rispetto degli impegni europei è stato uno degli elementi di riferimento delle indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria.

di cui ho delineato i tratti principali per quel che riguarda le innovazioni introdotte nella Nota stessa. La manovra di bilancio articola i suoi effetti attraverso il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, il disegno di legge finanziaria, che è stato presentato, e un provvedimento di urgenza, in materia prevalentemente fiscale, che viene dichiarato collegato alla manovra. (ed è una parte significativa della Nota di aggiornamento), la Nota prevede che vengano collegati alla manovra anche altri testi normativi in corso di preparazione: il disegno di legge delega per il riordino dei tributi statali, il disegno di legge di revisione del Testo unico per gli enti locali, il disegno di legge delega sul federalismo fiscale, il disegno di legge sulla riorganizzazione e razionalizzazione degli apparati amministrativi, il disegno di legge sulle misure in materia di liberalizzazione, nonché il disegno di legge, già presentato, sui servizi pubblici locali. *(Richiami del Presidente).* Signor Presidente, concludo sottolineando che, sul fronte degli strumenti, la Nota di aggiornamento chiarisce una questione che era rimasta aperta nel DPEF: la mancanza di un'indicazione organica di tutti gli strumenti di attuazione, che oggi viene completata. Signor Presidente, ho terminato. Credo di aver svolto il compito, da un lato, di illustrare la Nota di aggiornamento e, dall'altro,

Signor Presidente, colleghi senatori e colleghe senatrici, la concisione e la stringatezza di un documento

Che questa mia affermazione sia suffragata non dai comportamenti dell'opposizione ma dai comportamenti

In particolare, in questa Nota di aggiornamento il Governo aveva dimenticato totalmente di fornirci i dati sul cosiddetto tendenziale. Se infatti si legge il documento a stampa che abbiamo di fronte, questa tabella non c'è; c'è soltanto quella relativa al quadro programmatico. Soltanto oggi e tardivamente, alla fine del dibattito, il Governo, accortosi di questa sua grave dimenticanza, ci propone il prospetto riguardante il bilancio tendenziale della pubblica amministrazione. Naturalmente, è chiaro che simili dimenticanze non sono assolutamente tali, ma è evidente che il Governo corregge, alla fine, con la fornitura del quadro tendenziale, alcune evidenti, evidentissime inesattezze che in questi mesi ha pronunciato e che, alfine, con il Documento di programmazione prima e con la Nota poi, sono state portate alla luce del sole. Cercherò di dire esattamente quali sono queste inesattezze.

le leggi in materia contabile le attribuiscono, vale a dire aggiornare i dati relativi al quadro macroeconomico e di finanza pubblica in relazione all'evoluzione degli andamenti. Di fatto, questa Nota interviene in misura significativa, i presupposti e gli obiettivi del prossimo esercizio finanziario contenuti nel DPEF di luglio, perché ben presto si sono dimostrati largamente inattendibili.

il quale sosteneva che il Governo Berlusconi aveva lasciato l'Italia allo sbando, allo sfascio, per scoprire poi che la crescita è andata un po' meglio, che le entrate sono aumentate e che il quadro economico

che questa insistenza, quasi drammatica e del tutto inattendibile, del Governo sulla presunta maggiore gravità della situazione di finanza pubblica odierna, addirittura rispetto a quella del 1992, ha creato nei mercati l'aspettativa di una manovra consistente nella quantità ed efficace nella struttura, sottoponendo il Paese ad un elevato rischio di declassamento del *rating* nel caso

lo dice la Nota, non lo affermiamo noi. Infatti, l'andamento particolarmente favorevole del fabbisogno, che segue un costante e crescente miglioramento rispetto allo scorso anno, costituisce la prova più evidente dell'efficacia delle misure poste in essere dal precedente Governo per garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nonostante una congiuntura che allora era meno favorevole di oggi.

Tale rapporto, che la Nota evidenzia, è addirittura inferiore a quello stimato prudentemente dal Governo Berlusconi in occasione dell'approvazione della legge finanziaria per il 2006 - che, ricordo all'Assemblea, dunque andava meglio di quanto avevamo prudenzialmente previsto - ed è di molto inferiore, soprattutto (ecco quell'allarmismo inutile e molto grave, di cui ho discusso poco fa) di cui ho discusso poco fa) a quello formulato dalla cosiddetta commissione Faini, che, ricorderemo, lo attestava al 4,6 per cento: un dato totalmente diverso da quello reale, minore di ben un punto rispetto a quello della famosa commissione Faini. Ciò ad ulteriore dimostrazione della correttezza dei dati previsivi formulati dal precedente Governo e della falsità della rappresentazione che veniva data dall'attuale Governo all'atto del suo insediamento. Non vi è dubbio che il miglioramento del fabbisogno (e qui la riconferma della nostra politica tributaria, oltre che economica) è attribuibile, quanto meno in parte, in parte significativa almeno, al positivo andamento del gettito che deriva dall'allargamento della base imponibile operato dal precedente Governo, pur in costanza di un abbassamento generalizzato delle aliquote nominali, cioè esattamente il contrario di quel che il Governo si accinge a fare.

convintamente contro questa Nota di aggiornamento al DPEF. Ribadisco: le considerazioni fatte solo parzialmente danno ragione del nostro voto contrario, che si rivela particolarmente convinto e significativo.

senatore Azzollini vi siano, sì, elementi di novità nella trasmissione dei dati del Governo, soprattutto per quanto riguarda il tendenziale; propongo tuttavia una questione sospensiva per poter valutare questi dati, alla luce degli ultimi elementi emersi.

e soprattutto, attraverso la Presidenza, all'attenzione della Giunta per il Regolamento, una questione che incide ed è il caso, perché si tratta di una questione incidentale - sui nostri lavori in maniera contraddittoria rispetto alle previsioni del Regolamento. Signor Presidente, so che qui in Senato prassi costante è quella che un collega senatore, subito dopo l'intervento dei relatori, in questo caso di maggioranza e di minoranza, possa proporre una questione sospensiva e, in altri casi, anche una pregiudiziale di costituzionalità. So che è prassi del Senato (secondo un'interpretazione devo ritenere abbastanza vicina allo spirito e alla lettera della norma, quindi pienamente giustificata) che si debba procedere immediatamente alla votazione. Se non che, signor Presidente, mi consenta di segnalare la necessità di una riflessione su questa previsione, perché in altra parte del Regolamento è tassativamente, anzi direi rigorosamente ed esplicitamente previsto che è impedito all'Assemblea di esaminare qualsiasi oggetto che non sia stato previsto nell'ordine del giorno dei nostri lavori. Anche qui, signor Presidente, la previsione letterale e dello spirito della norma è chiarissima: non si può discutere in Assemblea di alcun oggetto che non sia previsto all'ordine del giorno. Signor Presidente, per l'inclusione di qualsiasi oggetto all'ordine del giorno, il Regolamento prevede esplicitamente le procedure che bisogna osservare.

Quindi, tutte le fattispecie per includere qualsiasi argomento all'ordine del giorno sono esplicitamente disciplinate dal Regolamento. Questo avvalora la norma principale, generale e, direi, di principio, signor Presidente, secondo cui non è possibile discutere in Assemblea di alcun argomento che non sia all'ordine del giorno. Mi deve consentire, non è tanto una questione formale e regolamentare, ma di tutela del diritto del senatore a sapere cosa si discute e, soprattutto, cosa è chiamato a votare.

il processo della manovra finanziaria. Apprezzo, quindi, perfino la responsabilità del collega Polledri, però, signor Presidente, non è possibile che un senatore - e tanto più il collegio dei senatori, cioè l'Assemblea

Signor Presidente, è una cosa assurda e che ritengo in contrasto con una norma esplicita del Regolamento. Tuttavia, ella mi dirà che il Regolamento prevede questa fattispecie. Signor Presidente, chiedo che la Giunta per il Regolamento, anche mettendo in discussione la prassi seguita attualmente, emetta un giudizio sul primato della fonte:

rispetto alla norma che prevede invece la possibilità di proporre all'improvviso una questione sospensiva o pregiudiziale.

da un punto di vista del ragionamento, ha pure un certo valore. Lei sa che alla Camera dei deputati, per poter porre una questione pregiudiziale o sospensiva prima dell'inizio della discussione generale, vi è l'obbligo di darne annunzio alla Conferenza dei Capigruppo, cioè vi è comunque la previsione che tale eventualità venga inclusa e annunziata per l'ordine del giorno. Infatti, quando si forma l'ordine del giorno, correttamente il Presidente della Camera lo prevede: «salvo eventuali questioni pregiudiziali o sospensive». anche che, se si vuole proporre una questione pregiudiziale o sospensiva successivamente, deve essere preventivamente presentata, in maniera che possa essere esplicitamente inclusa nell'ordine del giorno.

da parte della Giunta per il Regolamento, affinché esamini se tra le due previsioni del Regolamento ve ne sia una che riconosce il diritto soggettivo del senatore e dell'Assemblea a sapere che cosa succede

al DPEF, stampata ufficialmente dal Senato della Repubblica, è un falso in atto pubblico, perché mancano gli andamenti tendenziali. Solo alle 19 di oggi pomeriggio,

L'argomento è molto semplice ed occuperà pochi secondi. Si tratta di questo: lei sa, signor Presidente, che il Documento di programmazione economico-finanziaria e, di conseguenza, un'eventuale Nota di aggiornamento allo stesso debbono essere discussi debbono essere discussi contestualmente da Camera e Senato, in sostanziale contemporaneità, anche se la contemporaneità non è naturalmente assoluta. Questo perché, essendo la Nota di aggiornamento un documento identico, per valore di indirizzo, al Documento di programmazione economico-finanziaria ed essendo questi due Documenti propedeutici alla definizione della legge di bilancio e della legge finanziaria, le risoluzioni che Camera e Senato approvano sulla Nota di aggiornamento, così come sul DPEF, possono essere distinte in qualche aspetto, ma debbono contenere sostanzialmente lo stesso indirizzo. In un sistema di bicameralismo perfetto come quello nel quale ci troviamo, infatti, il Governo non saprebbe quale di due risoluzioni diverse, o formulate in tempi clamorosamente diversi, dovrebbe seguire nella definizione dei documenti di bilancio. Ora, signor Presidente, il relatore non ha sottolineato un aspetto, anche per non mettere in evidenza una qualche incongruenza del nostro modo di procedere: la Nota di aggiornamento, che stiamo discutendo, alla Camera è già stata discussa e ha già dato luogo all'approvazione della relativa risoluzione. Al Senato la proposta di risoluzione, per quello che concerne la maggioranza (ma credo che questo riguarderà anche la risoluzione dell'opposizione), è sostanzialmente stata presentata in termini identici a quella presentata dalla maggioranza alla Camera. La proposta di non procedere neppure oggi, quando già il Senato ha accumulato un ritardo, alla discussione sulla Nota di aggiornamento, è contraddittoria con questa finalità, a cui risponde la Nota di aggiornamento stessa. Anche solo un giorno ulteriore di tempo recherebbe un danno, a mio giudizio, giudizio, alla credibilità del Senato, come sede nella quale si forma un atto di indirizzo verso il Governo che abbia la stessa forza dell'analogo, anzi identico, atto di indirizzo che viene approvato

attraverso l'esposizione della sua relazione, che il Governo fosse più puntuale nella presentazione degli andamenti tendenziali, in particolare per quanto riguarda il rapporto *deficit*-PIL. In quella sede, cioè la scorsa settimana,

il tendenziale relativo al rapporto *deficit*-PIL. Questo è avvenuto nella giornata di oggi, signor Presidente, perché così abbiamo deciso in Commissione, così il Governo si era impegnato a fare e così è stata l'organizzazione dei nostri lavori. Se la Commissione avesse avuto la possibilità di riunirsi prima,

al Senato si fanno delle cose e alla Camera se ne fanno delle altre, pur salvaguardando l'autonomia dei due rami del Parlamento vi è l'esigenza che oggi si proceda, perché non credo che non vi sia la possibilità di procedere con i nostri lavori. Concludo, signor Presidente, ricordando che la richiesta di avere delle valutazioni più rispondenti rispetto agli andamenti tendenziali non solo è stata formulata dal relatore, ma è stata formulata da tutti i senatori che sono intervenuti nel dibattito in Commissione, sia di maggioranza che di opposizione. Quindi, di questo problema vi era ben coscienza rispetto al dibattito che abbiamo svolto; un problema che si è risolto oggi attraverso la presentazione

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi associo alle motivazioni che sono già state illustrate da parte del presidente Morando e del collega Ripamonti in ordine al fatto che non vi sono ragioni per rallentare la procedura che è in corso di perfezionamento e per licenziare una Nota di aggiornamento al DPEF che comunque appare rilevante, appunto, per gli indirizzi necessari nella politica economica del Governo. Come ha ben ricordato il collega Ripamonti, la Commissione ha approfondito ogni aspetto della Nota di aggiornamento presentata, ha preso atto delle precisazioni e delle integrazioni presentate dal Governo, oggi illustrate dal Sottosegretario alla Commissione in modo sicuramente non sintetico ma ampiamente esaustivo, ne hanno preso atto tutti i componenti presenti e partecipanti ai lavori. La Camera ha già realizzato questo passaggio, particolarmente importante e delicato, visto anche il prosieguo dei lavori cui siamo chiamati sulla legge finanziaria che dovremo andare ad esaminare e votare prima della fine dell'anno; credo lo si debba consentire anche qui, visto che non ci sono assolutamente ragioni, né di opportunità, né di soddisfazione delle giuste pretese che gli onorevoli colleghi potrebbero avanzare di avere tutte le informazioni al riguardo, avuto presente che le stesse sono state date, e quindi chi avesse voluto approfondire ogni aspetto aveva il luogo, la possibilità e il tempo di farlo.

finanziarie che si sono verificate nell'ultimo periodo: mi riferisco in particolare al tema delle maggiori entrate fiscali e alla sentenza dell'Unione Europea in materia di detraibilità dell'IVA. Non vedo motivi per cui il Senato non possa adempiere a quello che è un suo dovere istituzionale. Per tali ragioni, il Gruppo Per le Autonomie ritiene che sia assolutamente priva di fondamento la richiesta di sospendere il dibattito in corso e la votazione prevista su questo argomento.

recuperate attraverso un passaggio da detrazione a deduzione. A questo punto cosa possiamo fare, se non chiedere un approfondimento di una Nota di aggiornamento che, ripetiamo, è troppo confusa, troppo

Ministro Mastella, ha tenuto l'Aula impegnata per tanto tempo, adesso contribuisca ai nostri lavori. Il

il rito odierno sulla Nota di aggiornamento del DPEF 2007-2011 non può essere consumato senza apportare elementi di verità, anche rispetto alla relazione del senatore Morgando, come ha sottolineato anche il senatore Azzollini. Questa Nota, pur lacunosa, omissiva e reticente sui saldi finanziari per gli effetti della sentenza europea sulla detraibilità dell'IVA, che voi avete sterilizzato negli esiti con il recente decreto, e sul debito per la riclassificazione dei debiti sanitari, è la dimostrazione della contraddittorietà della politica economica perseguita dal Governo Prodi, certificata peraltro della presentazione della legge finanziaria dentro una manovra di bilancio che presenta un pericoloso scostamento dalla risoluzione approvata dal Parlamento. Prende atto del buon andamento delle entrate, smentendo l'ipotesi della pesante eredità sui conti pubblici. La finanziaria non è figlia del Documento di programmazione economico-finanziaria La correzione dei conti pubblici viene affidata in larga misura all'entrata, anziché ad una compressione strutturale della spesa. Gli sprechi aumentano anziché diminuire. Si aggrava il *deficit* infrastrutturale del Paese per l'incapacità di affrontare le grandi scelte europee, a cominciare dalla direttrice Torino-Lione. Non si affronta il problema dell'evasione fiscale attraverso lo strumento principe del contrasto di interesse! Si complica la vita dei cittadini contribuenti, costretti a nuovi, onerosi e complicati adempimenti tributari. La drammatizzazione dei conti pubblici ha rappresentato un alibi per operare una forzosa e sbagliata redistribuzione del reddito, da una parte, e la creazione di fondi e fondini per soddisfare le clientele, gli apparati e i parassitismi. Questa legge finanziaria è già tutta una gigantesca, abbondante mancia. Non avete combattuto gli sprechi degli enti locali, né burocrazie elefantiache. Avete preferito la via facile di maggiore tassazione diretta e di fiscalità locale aggiuntiva, come nel caso dell'ICI, smentendo gli stessi vostri impegni. Su questo punto, in particolare, avete mentito clamorosamente al Parlamento, nel momento più alto, quello che fissa le linee di programmazione finanziaria. Dovreste coerentemente aggiornare la risoluzione Finocchiaro, se non volete che questo Documento passi per un falso in atto pubblico. Non è solo il rapporto manovra sull'entrata rispetto alla spesa ad essere alterato profondamente. Avete espropriato il TFR dei lavoratori barattandolo con colpevoli connivenze di tanti distratti, con la «rottamazione» dei lavoratori cinquantenni. È una manovra che non contraddice solo i vostri impegni. Questa legge finanziaria, nata sull'asse Prodi-Rifondazione-Epifani, è il frutto dell'originale alleanza fra oligarchie finanziarie e lotta di classe; una finanziaria che opera una sedicente redistribuzione del reddito alimentando il conflitto sociale, anziché favorire una vera, autentica redistribuzione e conseguente mobilità sociale nella crescita economica e nello sviluppo complessivo del Paese. E' profondamente sbagliata nell'impostazione, eccessiva nella dimensione, insufficiente nella qualità, rischiosa negli interventi, priva di riforme strutturali, pregiudicando le possibilità di crescita del Paese. Manca una seria lotta agli sprechi; un ridimensionamento della spesa pubblica, partendo da una seria lotta agli sprechi, da una riduzione dell'effimero istituzionale (di cui simbolo é il veltronismo), delle missioni intercontinentali, del turismo assessorile, delle aperture di ambasciate newyorkesi (invece di pensare a risolvere il drammatico problema dei rifiuti in della convegnomania, sostenuta attraverso la disponibilità delle aziende municipalizzate e di *public utilities*. Colpite pesantemente il bene casa e la famiglia nel passaggio generazionale, ripristinando la tassa di successione. Si accrescono le burocrazie e gli adempimenti anziché semplificare e favorire i contribuenti. La prossima dichiarazione dei redditi, altro che lunare, sarà galattica! Questa decisione di bilancio che, forse, potrà salvare gli equilibri sinistri della maggioranza con l'affermazione del principio del «tutto e subito» e di una finanziaria ideologica, classista, antagonista dei ceti medi produttivi, facendo l'opposto del necessario, dunque non è solo un'occasione mancata ma un serio ostacolo allo sviluppo del Paese. Purtroppo, signor Presidente, per migliorare questa manovra di bilancio non basta un gruppo di volenterosi, una vasta schiera di uomini liberi e forti, capaci di assumersi, con coraggio, responsabilità per il bene comune fuori dalle appartenenze e da ogni vincolo.

e pone un problema del tutto inedito di compatibilità con le procedure parlamentari previste dalla sessione di bilancio. La lettera in oggetto specifica che si tratta di un testo di 300 pagine di articolato con minuziose modifiche ordinamentali, che in alcuni settori sono, nei fatti, incompatibili con i tempi rigorosamente scanditi e contigentati della sessione di bilancio. La lettera, che facciamo nostra, aggiunge che la natura prevalentemente ordinamentale ed estremamente analitica del testo toglie ogni giustificazione al vero e proprio esproprio delle competenze delle Commissioni di merito da parte della Commissione bilancio, motivato solo se i fini sono essenzialmente e rigorosamente legati alla manovra economica e di finanza pubblica. Non a caso, la procedura di bilancio prevede, con la legge finanziaria, la possibilità di presentare uno o più provvedimenti ad essa collegati, cui si applicano, naturalmente, analoghe garanzie quanto ai tempi di approvazione e all'ammissibilità degli emendamenti.

di ciò che il Presidente dell'altro ramo del Parlamento riterrà di fare rispetto a questa richiesta, e di tenerne conto sin d'ora come di una richiesta del nostro Gruppo, affinché le prerogative parlamentari siano rispettate e la finanziaria non venga utilizzata come una legge *omnibus* in cui far entrare modifiche ordinamentali che nulla hanno a che fare con la manovra di finanza pubblica. Detto questo - e la ringrazio dell'attenzione - passo all'argomento del nostro dibattito. Il relatore di minoranza, ma anche altri colleghi intervenuti prima nel dibattito procedurale, hanno fatto presente come questa Nota di aggiornamento al DPEF sia probabilmente la più breve e la meno adeguata che si possa riscontrare negli ultimi decenni. C'è però, parere, una ragione politica di fondo che non nasce dall'incuria del Governo o dalla scarsa capacità tecnica del Ministro, che anzi è stimato ovunque proprio per le sue doti di esperto di finanza pubblica e per la sua esperienza pluriennale anche in istituzioni prestigiose come la Banca centrale europea, ma nasce da un problema politico centrale a cui questa Nota di aggiornamento non risponde e a cui la maggioranza e il Governo non rispondono. Siamo in presenza, intanto, di una situazione procedurale complessa, perché, nonostante quello che ha ricordato prima il presidente della Commissione, Morando, l'aver ottenuto soltanto oggi la tabella sugli andamenti tendenziali, su un documento che è stato trasmesso alla Presidenza il 30 settembre, cioè contestualmente alla legge finanziaria trasmessa quel giorno stesso alla Camera, in realtà è una trascuratezza, una manchevolezza del Governo che ha di fatto "disassato" le procedure tra la Camera e il Senato e ci ha posto in condizione di discutere oggi di qualcosa, la Nota di aggiornamento, che in realtà la legge finanziaria ha già trascurato e di cui la Nota di aggiornamento stessa non tiene assolutamente conto. Quando il Governo presentò il DPEF, nella lettera con cui il ministro Tommaso Padoa-Schioppa accompagnava il testo, parlando dei conti pubblici sottolineava il fatto che «la dimensione dello squilibrio» - con particolare riferimento evidentemente al debito «rende indispensabile intervenire anche su tendenze strutturali della spesa pubblica che sono sempre meno favorevoli, dunque sui quattro grandi comparti -sistema pensionistico, servizio sanitario, amministrazioni pubbliche, finanza degli enti decentrati che ne rappresentano circa l'80 per cento». Si annunciava, cioè, in questa lettera che sui quattro grandi comparti della spesa pubblica il Governo avrebbe proposto, attraverso la legge finanziaria, riforme con cui ridurre strutturalmente la spesa per poter risanare i conti senza dover dare luogo a maggiori entrate e ad un inasprimento fiscale. Ora, su questo impegno il Ministro ha speso tutta l'estate, ha rilasciato interviste ovunque e ha cercato di assicurare al Governo una credibilità riformatrice che in realtà, alla luce della finanziaria, vediamo non esistere, perché esattamente su quei quattro comparti che rappresentano l'80 per cento della spesa pubblica non una misura di riforma è contenuta nella finanziaria, ma solo misure di aumento delle entrate di vario tipo che rovesciano totalmente quell'impostazione. È vero che la Nota di aggiornamento fa riferimento alla differenza del quadro macroeconomico, ma ci si sarebbe aspettati in qualche misura misura un cambiamento radicale di linea politica, quello per cui si sono annunciati a giugno e sono stati fatti votare da quest'Aula e dall'Aula della Camera un Documento di politica economica, una strategia di politica economica che guardava in direzione delle riforme, che si è trasformato invece, nel momento in cui il Governo ha emanato le disposizioni normative, nel suo contrario, cioè nel mantenimento assoluto dello *statu quo* per quel che riguarda i comparti di spesa, e nell'innalzamento della pressione fiscale a livelli di *record*. Occorrerebbe molto più tempo di quello che abbiamo a disposizione per rendere conto di questo cambiamento di strategia. Voglio dare solo qualche indicazione e qualche numero ai colleghi. di legge finanziaria, nonostante il Governo si fosse impegnato e avesse detto in campagna elettorale che non avrebbe inasprito la pressione fiscale né introdotto nuove tasse, ci sono ben 67 tasse che sono state o inasprite o introdotte *ex novo*. Qui ne abbiamo un elenco dettagliato, tra il decreto-legge che arriverà presto al nostro esame, la legge finanziaria e l'unico documento collegato fino ad adesso disponibile, cioè la legge delega in materia fiscale. Non solo, la stima che è stata fatta sulla base dei conti la dice lunga di come il Governo abbia rinunciato a qualunque azione di riforma. Infatti, il complesso della manovra, di circa 35 miliardi, è garantito per quasi l'85 per cento da entrate aggiuntive e solo per il 15 per cento da rimodulazioni di spesa. Gli scenari di oggi prevedono che i 35 miliardi ricadranno tutti sui cittadini e sul sistema produttivo e nulla ricadrà, invece, sulla qualità e sulla quantità della spesa della pubblica amministrazione. Sempre per dare qualche numero, potremmo elencare quali sono i principali incrementi fiscali; ma questo lo vedremo. La politica ma questo lo vedremo. La politica fiscale è stata presentata come una svolta in direzione dell'equità e del riequilibrio, per cui chi più ha paga in percentuali superiori rispetto a prima e chi meno ha dovrebbe essere alleviato dal punto di vista fiscale. Si è detto che anzi, revocando il secondo modulo della riforma Tremonti, si restituiva a chi aveva avuto minori vantaggi, cioè i meno abbienti, e si riprendeva da chi aveva avuto

arrivava fino a 15.000 euro di reddito lordo annuo e oggi si attesta a 7.500 euro - ma che la nuova curva di aliquote e scaglioni fa sì che sì che gli inasprimenti fiscali partano dai 20.000 euro. Non credo che sia rispettato quello *slogan* che una componente della maggioranza aveva lanciato: «Anche i ricchi piangano». Qui piangono - e moltissimo - anche quelli che sono molto meno ricchi, o addirittura poveri. Per non parlare di ciò che avviene per quanto riguarda, per esempio, il lavoro a tempo determinato. Con questa finanziaria, per tutti coloro i quali abbiano un contratto in qualche modo a tempo determinato, un contratto di lavoro flessibile, per i quali la maggioranza in campagna elettorale si è stracciata le vesti promettendo che, se avesse vinto, avrebbero avuto vantaggi straordinari e sarebbero usciti dal limbo della precarietà nel quale il Governo Berlusconi, colpevolmente e senza alcuna sensibilità sociale, li aveva cacciati, ebbene, per i collaboratori a progetto, per i collaboratori a termine l'innalzamento delle aliquote previdenziali azzera totalmente l'eventuale beneficio fiscale e complessivamente diminuisce la busta paga degli stessi. Faccio un esempio soltanto: un collaboratore che non abbia nessun familiare a carico e che abbia una retribuzione lorda annua di 20.000 euro vedrà ridurre, in virtù dell'aumento dei contributi previdenziali, il suo compenso lordo di 162 euro all'anno; credo che sia un bel regalo in difesa di questi lavoratori! Un parasubordinato che abbia moglie e figli a carico dovrà lasciare alla difesa dei più deboli - che non si capisce a questo punto chi siano - 77 euro sul campo. Proprio l'innalzamento delle aliquote contributive provoca questi effetti su tali redditi. Ma non solo, ne provoca di maggiori. Chiunque abbia un minimo di contatto con il mondo delle imprese, e soprattutto col mondo delle piccole e medie imprese che si sono avvalse delle forme di lavoro flessibile per introdurre nel mercato del lavoro nuove persone che prima non lavoravano, di varia età che noi abbiamo contratti flessibili che si sono applicati ai giovani, ma abbiamo anche contratti flessibili che si sono potuti applicare a persone che altrimenti sarebbero state fuori dal mercato del lavoro),

ha ingannato per tutta la campagna elettorale, strappandone probabilmente il voto, e vincendo le elezioni per 24.000 voti, quindi con il voto determinante anche di questi giovani e di queste persone. Ebbene, grazie alla grazie alla finanziaria che spero cambi (e spero cambi grazie al nostro lavoro), costoro si vedranno, non soltanto penalizzati se manterranno il loro contratto, ma espulsi dal mercato del lavoro. Complimenti, complimenti soprattutto a quei colleghi dell'estrema sinistra che hanno messo i lavoratori al centro della loro attenzione! I lavoratori ringraziano e vorrebbero che l'attenzione fosse distolta a favore di altri, ma possiamo andare avanti su tutto. In realtà, la filosofia con cui il Governo ha proceduto, e di cui nella Nota di aggiornamento non vi è traccia

accade, ritiene che l'economia sia statica e ritiene di poter andare a prendere risorse per lo Stato da quelli che sono i beni individuabili, i beni registrati, i beni immobili, le posizioni che sono misurabili, indipendentemente dagli effetti che questo produrrà sull'economia.

Presidente, diventa abbastanza facile portare la discussione dalla Nota di aggiornamento ai contenuti e alle misure previste

ad esporre due o tre questioni che ritengo importanti circa la Nota di aggiornamento, rinviando ovviamente la discussione sulla legge finanziaria a quando saremo investiti di questo provvedimento. Intanto, la Nota sancisce due novità che si sono verificate nell'economia italiana e sull'andamento dei conti pubblici nel 2006, una positiva e l'altra un po' meno positiva: quella relativa al miglior andamento delle entrate e quella relativa alla sentenza della Corte di giustizia europea sulla detraibilità dell'IVA. Vanno evidenziate queste due questioni, in particolare partendo dal fatto che, fortunatamente, c'è sul 2006 una crescita del prodotto interno lordo leggermente superiore rispetto alle previsioni: si passa all'1,5-1,6 per cento, mentre le prime previsioni indicavano l'1,3 per cento. Quindi, c'è un andamento del prodotto interno lordo migliore del previsto e questo prevedere un miglioramento delle entrate tributarie, conteggiate, dal punto di vista strutturale, per 6 miliardi di euro.

Probabilmente iniziano a funzionare alcune misure adottate nella scorsa finanziaria che restringono l'andamento della spesa sul 2006. È un'ipotesi. Ritengo che il Governo avrebbe dovuto essere più preciso al riguardo.

Questo dato risulta in modo chiaro dalla tabella che il Governo ha presentato circa gli andamenti tendenziali.

Augurandoci che le previsioni si avverino, questo è dovuto al fatto che il debito diminuisce e ciò avviene anche perché si riesce ad invertire la tendenza riguardante l'avanzo primario, che dovrebbe cominciare a riprendere un ciclo positivo. Ricordo che l'impatto della sentenza della Corte di giustizia europea sulla indetraibilità dell'IVA produce un *deficit* del 4,8

Ovviamente l'opposizione porta a dimostrazione di questa sua affermazione il fatto che il *deficit* risulta migliore delle previsioni. Voglio sottolineare a tale riguardo - l'ho già fatto in Commissione e voglio ricordarlo sommessamente in Aula - che il dato rilevante ai fini dell'andamento dei conti pubblici per il nostro Paese non è tanto l'andamento del *deficit*,

per gli interessi sul debito, e l'avanzo primario. Voglio ricordare anche che la situazione economica del nostro Paese si caratterizza, a differenza di quanto avviene negli altri Paesi, nostri competitori diretti, anche per altri elementi che sarebbe opportuno ricordare. Forse anche questi denotano una situazione difficile che si richiama rispetto alla situazione nel 1992. Abbiamo perso in questi anni quote rilevanti sui mercati internazionali; aumento della produttività nel nostro Paese, ma inferiore rispetto agli altri Paesi, nostri competitori diretti, mi riferisco in particolare alla Francia ed alla Germania; infine,

recentemente e come affermano anche noti economisti, cosiddetti indipendenti, che sarebbe stata necessaria solo una manovra finanziaria di aggiustamento dei conti pubblici e per il resto lasciare fare i mercati? Credo di no. Se l'economia

Ed è questa una delle misure che abbiamo inserito nella finanziaria. Ma vi è un aspetto rilevantissimo che va posto all'attenzione della nostra discussione: abbiamo una eredità più pesante del previsto.

Se si può parlare di vendetta, è la vendetta della ex maggioranza, che ha bruciato i ponti mentre scappava e ci ha lasciato una situazione in cui non vi era più la possibilità di intervenire sulle misure

è un po' pessimista riguardo al passato. Però, in queste ore vi è un interrogativo di fondo: ma la trasmissione de «Le Iene» trasmetterà

che aveva promesso felicità a tutti gli italiani. Pertanto, questa situazione di felicità è contagiosa; una condizione di assenza di dolore.

data, la commissione Faini, che lamentava sfracelli, addirittura parlava di un rapporto *deficit*-PIL al 4,6

e gli italiani cominciano a vedere chi fa uso di certe sostanze. Si era anche detto che non si sarebbero messe le mani nelle tasche dei lavoratori, ma il TFR di chi è?

questo è un taglio di spesa? A casa mia è un aumento di entrate. Se possiamo permetterci di consegnare un giudizio agli italiani che hanno la ventura di ascoltarci, crediamo sia una cosa ingiusta.

2-3 miliardi non di tagli di spesa, ma di minori trasferimenti agli enti locali. Pensiamo forse che non faranno pagare niente ai cittadini?

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, presidente Prodi e il ministro Padoa-Schioppa hanno dovuto ammettere che il buco nei conti pubblici non c'era e che hanno ereditato una situazione finanziaria in linea con gli impegni presi in sede ECOFIN nel luglio 2005. Sia il Governo che il relatore di maggioranza Morgando dell'Ulivo hanno riconosciuto che nel corso del 2006 ci sono state maggiori entrate per 6 miliardi di euro rispetto alle catastrofiche previsioni fatte nel luglio scorso con il DPEF e che dette entrate sono a carattere strutturale, tanto da prevedere maggiori entrate anche nel 2007 per 5 miliardi. Non solo i caratteri regolativi della finanziaria dell'anno scorso hanno dato stabilità al quadro del prelevamento delle risorse, ma hanno prodotto i propri effetti anche sul lato della spesa,

il fabbisogno nel settore statale è sceso da 69 miliardi a 44 miliardi di euro, diminuendo di ben 24 miliardi di euro. Nel giugno scorso avete messo in piedi la famosa commissione Faini che non solo è costata soldi, ma ha sbagliato ogni previsione e vi ha fatto fare una pessima figura.

a causa della paura che avete ingenerato negli investitori istituzionali per il rischio Italia. I danni delle previsioni al ribasso del DPEF di luglio, della indetraibilità dell'IVA sugli immobili della prima versione del decreto Visco-Bersani e delle imprudenti dichiarazioni di Prodi sulla situazione Telecom sono stati tutti registrati con forti impatti negativi sui mercati finanziari, pregiudicando la credibilità dei nostri conti pubblici e dei fondamentali del nostro sistema di finanza privata. Come si sarebbe detto nei tempi andati: «dilettanti allo sbaraglio». Tornando alla Nota di aggiornamento, così com'è stato rilevato dal Servizio bilancio del Senato e dallo stesso relatore di maggioranza, essa manca di un quadro degli andamenti tendenziali ed anche di un quadro programmatico che fornisca il dettaglio dei principali aggregati di spesa. Manca inoltre un quadro del mutato fabbisogno, sia tendenziale che programmatico, che tenga conto anche dell'impatto che eserciteranno i rimborsi IVA sulle automobili d'azienda, che verranno chiesti dai contribuenti in virtù della ben nota sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea. Se è fondata la stima di 3.700.000.000 di euro di minor gettito per il 2006 e il pagamento di 13.400.000.000 di euro per il rimborso degli arretrati relativi agli anni 2003‑2005, vogliamo capire come si spalma questo nuovo debito negli esercizi successivi al 2006, se ci saranno scaglionamenti e con quali interessi. Vogliamo anche capire come inciderà sul debito pubblico la minaccia dell'Eurostat indirizzata all'ISTAT e pubblicata dall'agenzia Reuters il 18 settembre scorso, secondo cui le cartolarizzazioni dei debiti sanitari verrebbero considerate non già una ristrutturazione del debito sanitario di alcune Regioni per pagare i crediti di privati, ma potrebbero essere considerate - secondo i parametri di Maastricht - dei veri e propri debiti pubblici. Secondo «Il Sole 24 ORE» del 20 maggio scorso, la stima di detto debito si aggira intorno a 12-15 miliardi di euro, con riferimento soprattutto alle Regioni Lazio, Campania ed Abruzzo. Vorremmo capire se la riduzione di due punti di PIL della Nota rispetto al debito indicato dal DPEF di luglio, che ingloba la riclassificazione delle operazioni di cartolarizzazione dei debiti sanitari, ignora la minaccia dell'Eurostat richiamata. Nulla viene detto al riguardo e a noi appare imprudente scontare una riduzione del debito sulla base di una riclassificazione che avviene in uno scenario a tinte fosche. La Nota fissa nuovi obiettivi di finanza pubblica, scontando maggiori entrate e minori spese in corso d'anno, ma non spiega - come detto - come saranno impiegati i migliori risultati di gestione. La finanziaria 2007, in discussione alla Camera, è uno strumento, oltre al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, per raggiungere tali obiettivi, tra cui il risanamento, lo sviluppo e l'equità. Nella finanziaria sono spariti interventi previsti dal DPEF del luglio scorso, come la riforma della previdenza, del pubblico impiego e della pubblica amministrazione, degli enti locali e della sanità; né si cita in Nota alcunché. Tutto viene rimandato a successivi provvedimenti, i cui effetti sulla finanza pubblica non sono però cifrati. Siccome il tema della famiglia è prioritario per l'UDC, perché esso è la sintesi di tutte le politiche di sviluppo e di equità sociale, ci permettiamo di invocare il Governo perché vada oltre gli articoli 4 e 192 della finanziaria 2007, ossia vada oltre il miliardo e 400 milioni di euro destinati agli assegni familiari, perché destinati solo ai lavoratori dipendenti, ignorando i lavoratori autonomi e i disoccupati, e vada oltre anche i 215 milioni di euro destinati a commissioni e consulenze per il Ministro per le politiche per la famiglia, per destinarli a politiche strutturali a favore della maternità e della donna madre che lavora, come asili nido (di cui nessuno più parla), tempi di pausa e di lavoro della donna lavoratrice, permessi retribuiti per la genitorialità. Vogliamo un'equità sociale vera, non di facciata. Vogliamo una finanziaria dove nessuno pianga, soprattutto i figli delle famiglie numerose italiane. intervengo sulla Nota di aggiornamento del DPEF relativo alla manovra di finanza pubblica 2007-2011 con una considerazione preliminare. Prendiamo atto che nella Nota di aggiornamento il Governo tiene conto del più favorevole andamento delle entrate e delle stime di crescita, di cui si è venuti a conoscenza dopo l'approvazione della risoluzione sul DPEF del luglio scorso. La Nota di aggiornamento pertanto - questa è la nostra considerazione preliminare - delinea una strategia più equilibrata rispetto al DPEF, in relazione all'obiettivo politico di un simultaneo raggiungimento delle finalità di risanamento contestualmente a quelle di sviluppo e di equità sociale. Farò riferimento più avanti a qualche cifra positiva sull'andamento della domanda interna e delle

Se questa considerazione preliminare è vera, va detto allora che erano assolutamente fondate le preoccupazioni che il nostro Gruppo (Rifondazione Comunista-Sinistra Europea) aveva posto sul DPEF, sia in sede di Governo che nel dibattito parlamentare, cioè che un'eccessiva adesione passiva ai parametri di Maastricht ed al Patto di stabilità ed un'enfatizzazione forse eccessiva della situazione dei conti pubblici non facessero prendere in considerazione una diversa impostazione macroeconomica. Tale impostazione - sostenuta da diversi economisti, con un appello importante, tra cui quello del professor Graziani - consiste in un'operazione tesa alla stabilizzazione del debito, ovviamente, soddisfacendo il vincolo europeo relativo al *deficit* e ricostruendo l'avanzo primario, per consentire realmente il rilancio di politiche di equità e di sviluppo. Sia chiaro: su questo aspetto è nostra opinione che la proiezione sul 2007 del maggior gettito emerso nel 2006, stimato nella Nota prudenzialmente in 5 miliardi (come dato strutturale), sia eccessivamente prudente, forse perché si poteva prevedere un'ulteriore riduzione dell'entità della manovra necessaria a raggiungere gli obiettivi del DPEF. Ma, nel contempo, mi sembra del tutto evidente che i dati del nuovo quadro degli andamenti tendenziali, di cui ci ha informato oggi il Governo con il sottosegretario Casula, forniscono un quadro sicuramente sotto controllo, diversamente da ciò che diceva il senatore Azzollini, confermando che il miglioramento non è dovuto al caso; è dovuto certamente ad un clima positivo e soprattutto al fatto, che alcuni considerano assolutamente negativo, che si è aperta una politica di riequilibrio dei pesi dei problemi del Paese, una politica che con chiarezza sta perseguendo una strada di lotta all'evasione e all'elusione fiscale e di nessuna apertura ai condoni. quindi, consapevole del fatto che nessuno può dire che questo miglioramento sia della domanda interna sia delle entrate è esclusivamente merito di questo Governo, ma certamente è il prodotto di un clima nel quale ognuno sta cercando di rapportarsi alla nuova situazione.

in realtà avrebbero permesso, a nostro avviso, una maggiore caratterizzazione della manovra sui diritti sociali e quindi una manovra che lasciasse qualche margine in più. Sia chiaro: la nostra è una critica costruttiva per contribuire a formulare una nuova strategia macroeconomica

superando ad esempio i *ticket* e i tagli agli enti locali non con pannicelli caldi (come mi sembra di apprendere da un incontro, avvenuto qualche ora fa, dei rappresentanti delle autonomie locali

affermi che il potenziamento della domanda interna, di cui la spesa sociale è alimentatrice, è un elemento che aiuta anche la crescita economica. Dopo di me il collega e compagno Albonetti dirà meglio, ma vorrei concludere con una considerazione sul tema dell'aumento della domanda interna che nel primo semestre 2006 si è realizzato e che è evidenziato anche nella Nota. L'aumento della spesa sociale, sia in termini di servizi ai cittadini sia in termini di misure di contrasto alla povertà, non solo è giusta, ma è fondamentale per aumentare la domanda interna. Le politiche liberiste che nel 2003 portarono all'interruzione, ad esempio, della sperimentazione di una misura di contrasto alla povertà come il reddito minimo di inserimento considerate - da un rapporto scientifico formulato da un comitato nominato peraltro dal ministro Maroni, quello del professor Ranci Ortigosa - politiche che, tra gli altri effetti, aumentavano la domanda interna.

è un punto in cui si annunciano i provvedimenti legislativi collegati. Noi del Gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea abbiamo letto con sorpresa che il Governo intende considerare come collegato anche il disegno di legge n. 772 sui servizi pubblici locali:

stiamo discutendo di un atto che è un falso in atto pubblico. Si tratta di un fatto formale, signor Presidente: ho qui la Nota di aggiornamento del DPEF che probabilmente tutti i colleghi hanno in mano in questa Nota formale non c'è il quadro tendenziale di finanza pubblica. Il quadro tendenziale di finanza pubblica,

non intestata al Governo, e con una tabella che dà il quadro tendenziale. Faccio notare però che le due cose, messe insieme, fanno formalmente del

in Commissione, che ancora io ho in mano come anonima, verrà incorporata in una Nota di aggiornamento-*bis* negli atti del Senato. Al di là di ciò, nella Nota ufficiale che presenta il quadro programmatico appare

ma sul falso in atto pubblico ci sono precedenti clamorosi da parte di questo Governo. Ricordo il decreto Visco-Bersani, che arrivò in quest'Aula con un provvedimento sull'IVA degli immobili che avrebbe dovuto incorporare una stima di oltre 15 miliardi di gettito. Era evidentemente un errore, ma per come era scritto e per come arrivò in quest'Aula era anche quello un documento falso. Al di là di ciò, signor Presidente, questa Nota di aggiornamento, così confusa e pasticciata, è in realtà piena, come dirò, di errori tecnici, che assumono valenza politica.

in ragione delle modifiche del quadro contabile o economico, che avvenivano dopo il DPEF di luglio. Quindi, essa si deve concentrare nella spiegazione di cosa c'è di diverso oggi rispetto al dato di luglio.

fatta da questo Governo, sia in termini di andamento dell'economia, che di finanza pubblica, è clamorosamente smentita dai dati ufficiali, che il Governo non ha potuto fare a meno di inserire nella Nota aggiuntiva, nascondendo i numeri, con un errore tecnico che assume valenza politica. Evidentemente Evidentemente il giochetto tra programmatico e tendenziale si associa al giochetto tra cassa e competenza; si confonde spesso il fabbisogno di cassa che alimenta che alimenta il debito pubblico con la competenza, che costituisce l'indebitamento netto valevole ai fini dell'Unione Europea, e - se mi permettete, cari colleghi, chi di voi ne sa ben più di me, che sono un semplice ragioniere - si confonde la differenza tra conto economico e stato patrimoniale. di mascheramento della realtà riguarda quanto il Governo intende fare con la finanziaria; manca l'anello di congiunzione tra il DPEF e la legge finanziaria. Vengo rapidamente alla Nota tecnica, che assume valenza politica.

mentre nel 2006 risulterebbe addirittura del 4,8 per cento, sia nella tabella che è stata inserita ufficialmente sotto il titolo programmatico sia in quella tendenziale. Qui c'è un errore tecnico, che andrebbe quantomeno corretto.

inglobando nell'anno 2006, sotto la voce «Indebitamento netto», l'intero debito pregresso di tutti gli anni passati.

politicamente fraudolenta, del fatto che i conti erano fuori controllo. Il trucco è nell'andamento del debito pubblico. Il debito pubblico, nella tabella fantasma, cioè nel dato tendenziale, caro collega di Rifondazione - e siamo tutti i giorni in Commissione insieme -, è già stabilizzato.

a nascondere il fatto che la correzione che la prossima finanziaria dovrà operare in termini di *deficit* pubblico è soltanto pari ad una cifra che oscilla tra i 13 e i 15 miliardi di euro. Questa è la parte di legge finanziaria che il Governo conferma, asserendo che dei 34,7 miliardi di euro di manovra complessiva, somma raggiunta ieri

che i 34 miliardi di euro derivano da 28 miliardi di maggiori entrate e da 6,7 miliardi di contenimenti di spesa, ne risulta che la legge finanziaria aumenta la spesa pubblica corrente di quasi 14 miliardi di euro. Ecco perché si mettono le mani in tasca ai cittadini; non ai cittadini ricchi, ma a quelli che avranno

trasferimenti, o a ridurre i servizi o ad aumentare il prelievo. Mi meraviglio che i sindaci possano accontentarsi del fumo negli occhi

un'ultima considerazione. Di questi trucchi contabili, di questi imbrogli e della confusione tra conto economico e stato patrimoniale voglio darvi due esempi, uno clamoroso e uno piccolo ma significativo. primo concerne il TFR, rubato ai lavoratori e portato all'INPS. Il TFR è un atto di diritto privato, soldi dei lavoratori soldi dei lavoratori che sono presso le imprese. In ogni caso, qualcuno mi deve spiegare perché un debito delle imprese verso i lavoratori diventa un'entrata pubblica in questa finanziaria e in questo bilancio. Questo è un mistero, da quando fra Luca Pacioli inventò la partita doppia! Qualcuno deve spiegare come funziona il trucco per cui un debito delle imprese

Vorrei richiamare l'attenzione anche dei colleghi dell'opposizione, anzi, chiedo scusa, dell'ex opposizione e attuale maggioranza. Era un auspicio da parte mia, consentitemi la battuta.

che tende a non far capire al Parlamento e al Senato di cosa stiamo parlando; non farlo capire all'opposizione ma neanche all'interno della stessa maggioranza.

contro l'approvazione della Nota di aggiornamento, perché essa non chiarisce nulla rispetto alla situazione economica attuale e anzi peggiora i contenuti dello stesso Documento di programmazione economico-finanziaria così come era stato approvato prima dell'estate in quanto, nello stesso Documento, erano state previste quattro direttrici di intervento che non vengono rispettate assolutamente nell'attuale finanziaria; ricordiamo ai colleghi e ricordiamo per il resoconto che le direttrici erano la sanità, il pubblico impiego, gli enti locali e il sistema pensionistico. Di fatto, nella finanziaria troviamo soltanto un intervento nei confronti degli enti locali, che è uno scaricabarile, perché poi saranno gli enti locali a dover recuperare le risorse con un inasprimento della pressione fiscale. fiscale. La ripuntualizzazione, quindi, e la presentazione dei dati programmatici in una succinta tabella che fa un tutt'uno dei dati tendenziali del 2006 e dei dati programmatici per il 2007 non ci lascia capire alcunché. L'unico chiarimento che si vorrebbe dare è quello relativo alla necessità di reperire risorse per l'IVA, ma nelle note che ci ha fornito oggi lo stesso Governo - ed era uno dei motivi della questione sospensiva presentata poc'anzi - il

con riferimento al 2006, che questa necessaria risorsa è stata anticipata con emissioni di debito che garantiranno un livello del conto di tesoreria largamente eccedente il limite di legge in modo da fronteggiare i pagamenti per rimborsi già dal gennaio 2007. Ovvero, ci dovrebbe essere un aumento del debito pubblico nel 2006, ma non totale, perché si dice anche che, successivamente, è stata adottata un'ipotesi di scaglionamento del rimborso nel periodo 2007-2009. Questa è la scarsa chiarezza, non si capisce nulla; non si capisce se l'aumento del debito nel 2006 è finalizzato al recupero dei 13.400 milioni se è così, non si capisce perché poi si prevede uno scaglionamento dal 2007 al 2009. Questi sono dati che fanno ballare non un miliardo, ma ben 5, 6, 7 miliardi e allora non si capisce come questa Nota di aggiornamento possa essere propedeutica alla costruzione della finanziaria. E' una Nota di aggiornamento che noi non possiamo approvare. Questa è la finalità della proposta di risoluzione, quella di rendere chiaro al Parlamento, agli italiani e ai mercati che il Governo in questo momento sta giocando con le cifre. Come dicevamo in Commissione, come ribadivamo qui poc'anzi e come sottolineava il senatore Baldassarri, è una Nota assolutamente reticente, assolutamente confusa, che cerca di non far capire la reale situazione, che cerca di non far vedere che non c'è bisogno di intervenire così pesantemente sul debito pubblico,

dato seguito al rigore che era già stato anticipato con la finanziaria del 2005, talché il fabbisogno è diminuito. Ciò significa che la finanziaria che è stata costruita per

più reale, più conseguente, più trasparente rispetto alla reale situazione, che è ben migliore di quella che si costruisce, e lo sa benissimo il Governo, perché ha costruito una finanziaria che di fatto ha soltanto una

che il cuneo fiscale vale 20-30 volte di più del TFR, e poiché nella finanziaria è scritto che le due cifre sono equivalenti, non si capisce se è un TFR che è stato valutato in misura ben più larga rispetto a quello che è il suo reale ammontare, o se invece è il cuneo fiscale che dovrà essere maggiorato per una trattativa in corso di cui non sappiamo i contenuti. Il Governo sta operando soltanto un riscontro a partite di giro. Non dà agli enti locali mentre poi gli dà la possibilità di aumentare la pressione fiscale; riduce il cuneo e contemporaneamente lo fa pagare al TFR e aumenta la pressione fiscale. Il tutto con una tabella che è soltanto un enigma, che sembra quasi

nel corso di questi mesi che ci separano dal luglio scorso. La Nota di aggiornamento del DPEF registra invece mutamenti che ci sono stati; quelli che non sono avvenuti riguardano le fondamenta stesse del giudizio che abbiamo formulato a proposito di una possibile comparazione, in termini di gravità, tra la situazione di finanza pubblica di oggi e quella dei primi anni Vorrei ricordare al senatore Azzollini che quella comparazione è fondata su due elementi essenziali, di cui il primo riguarda le dimensioni dell'avanzo primario. Nella seconda metà degli anni Novanta, con uno sforzo eccezionale del Paese, si portò l'avanzo primario - tutti qui sanno di cosa si tratta

questo miglioramento dell'avanzo primario italiano «spettacolare». Lo chiamò proprio così: lo spettacolare risultato ottenuto dal Governo italiano in termini di miglioramento dell'avanzo primario. L'avanzo primario, che ancora nel 2001 per cento del prodotto interno lordo, nel 2006 è negativo, è cioè un disavanzo primario, come risulta dalla Nota di aggiornamento. Questo è il punto di assoluta gravità; il primo elemento del giudizio di gravità sulla situazione che noi registriamo e che la Nota di aggiornamento peggiora, perché tiene conto dei risultati di finanza pubblica indotti dalla sentenza sulla detraibilità

per la prima volta torna a crescere, e torna a crescere nei tendenziali in maniera significativa. Ecco perché noi diciamo che la situazione di finanza pubblica è assai grave, tanto più grave in quanto si accompagna ad un elemento che riguarda purtroppo l'economia reale. Ma a differenza di quello che accadeva nei primi anni Novanta, abbiamo una crescita del prodotto interno lordo da molti anni uguale o vicina allo zero e una situazione nella quale - ciò che è più preoccupante - la produttività totale dei fattori, cioè l'indice fondamentale della capacità di crescere del Paese nel medio e nel lungo periodo, addirittura decresce. Purtroppo, la Nota di aggiornamento non cambia nessuno di questi tre elementi di valutazione, anzi, come ho già detto, la stessa Nota, successivamente alla sentenza relativa all'IVA, è costretta a prendere atto di ulteriori peggioramenti.

Cominciamo da quello negativo. È già stato detto dal relatore e da molti altri che sono intervenuti in questo dibattito: si tratta delle conseguenze sul bilancio pubblico della sentenza della Corte dell'Aia sulla detraibilità dell'IVA.

peggiora, solo a causa di questa sentenza, dell'1,2 per cento del prodotto interno lordo. Signor Presidente, richiamo l'attenzione di tutti, in particolare del Governo (ho presentato infatti con il senatore D'Amico

non ha dimostrato che la sentenza avrebbe conseguenze finanziarie rilevanti sulla finanza pubblica italiana». Signor Presidente, se non è rilevante un 1,2 per cento di prodotto interno lordo, di peggioramento dell'indebitamento netto, cosa è rilevante? Chiedo al Governo di venire in Parlamento a riferire circa le responsabilità politiche, giuridiche e tecniche che hanno portato il Governo italiano a non essere in grado di dimostrare in sede di Corte dell'Aia ciò che questa Nota di aggiornamento - altro che non contare nulla!

fosse anche soltanto per il fatto che registra la novità, negativa, rappresentata dalla sentenza della Corte dell'Aia in materia di IVA. Le due novità positive, invece, sono quella relativa alla crescita del prodotto interno lordo, un po' più alta di quella prevista a luglio, e di quella prevista a luglio, e quella relativa alla crescita delle entrate, che crescono molto di più di quanto fosse previsto a luglio. Nell'anno in corso il prodotto interno lordo è previsto crescere dalla Nota di aggiornamento di un punto decimale in più rispetto a quello che era previsto a luglio. un punto decimale in più. Senatori dell'opposizione, vi prego, gli entusiasmi mi sembrano del tutto ingiustificati. Io invece voglio cogliere l'elemento positivo a cui ci sollecita questo dato. Senza troppo entusiasmo dobbiamo infatti chiederci: a che cosa si deve questo aumento del prodotto interno lordo, più elevato delle previsioni, anche se di poco, ma più elevato? Si deve alla domanda interna - qui non ci sono davvero ragioni di entusiasmo, perché rimane una domanda interna un poco migliore, ma assolutamente in chiave ancora molto bassa - e a - e a qualche piccolo segnale che viene dal mercato esterno, cioè dalle esportazioni. Ciò potrebbe voler dire, signor Presidente, che in questo momento abbiamo finalmente un apparato produttivo che negli anni duri e lunghi di crescita zero si è ristrutturato. Abbiamo pagato un prezzo in termini di quota di commercio mondiale in questa fase molto dura e molto lunga,

Perché richiamo questo elemento? Perché, se tutto questo fosse vero, e non è escluso che lo sia (lasciamo perdere questa diatriba ridicola sul merito - è mio, è tuo, c'era il Governo già fatto, no, è stata la faccia di questo Ministro

noi in una situazione nella quale l'apparato produttivo italiano, dopo lunghi anni di sofferenze e di ristrutturazione, si è rimesso in condizione di competere, è questo il momento delle riforme strutturali dal lato dell'offerta: liberalizzazioni, concorrenza dove non ce n'è, superamento dei mercati chiusi, infrastrutturazione materiale e immateriale del Paese. Se noi facessimo un salto da questo lato, allora questo apparato produttivo ristrutturato, per parte sua e senza grande contributo pubblico, potrebbe davvero far tornare l'Italia su posizioni di primato. Questa è la sfida aperta, questa è la riflessione che a mio avviso dovrebbe essere suggerita a tutti noi

la Nota di aggiornamento è incoraggiante esattamente per la ragione opposta a quella di cui ha parlato il collega Tecce, vale a dire perché contiene quell'elenco dei collegati.

che non solo non è destinata a ripetersi, ma addirittura nei prossimi anni - si sa come funziona questo meccanismo - produrrà una riduzione di gettito in rapporto alla rivalutazione dei beni di impresa effettuata sulla base di questa norma. In secondo luogo, abbiamo

mio giudizio si tratta di una stima realistica -, sottratto all'aumento complessivo che si sta determinando ciò che viene dalla norma sulle rivalutazioni dei beni di impresa e ciò che viene dal ciclo,

il Governo ha applicato un tasso di flessibilità delle entrate all'aumento del prodotto interno lordo del 2005 e non del 2006.

che non è perfettamente spiegato: il rapporto tradizionale tra miglioramento delle entrate e miglioramento del ciclo si sta modificando; il tasso di flessibilità è del tutto diverso e anomalo rispetto a

è un aumento delle entrate molto significativo - che la pressione fiscale 2006, cioè il rapporto tra tributi e contributi in rapporto al PIL, cresce vistosamente dello 0,8 per cento di PIL rispetto al 2005. rispetto al 2005. Ma se questo è vero, allora ci troviamo in presenza di un altro dato molto interessante. Sarebbe dimostrato che ci può essere un buon andamento della crescita anche in un contesto in cui la pressione fiscale aumenta di quasi un punto di PIL. Da questo bisognerebbe dedurre forse, signori dell'opposizione, che di per sé conta certo la quantità - la pressione fiscale aumentata deprime la crescita ma quando il contesto internazionale è positivo e la qualità dell'aumento delle entrate è di un certo tipo, forse questo aspetto depressivo è minore che in altri casi. Lo richiamo perché

dell'equità e dello sviluppo è certamente condivisibile, ma ad una condizione: siano posti degli aggettivi! Signor Presidente, svolgerò una breve replica su due punti che mi sembra siano stati oggetto di notevole attenzione nel corso del dibattito.

Ho l'impressione che qui vi sia un sacco di gente che ha poca memoria, perché ho provato ad andare a ricostruire quanto è successo negli anni precedenti.

fosse stata fatta notare questa carenza e fosse stato richiesto al Governo di fornire le informazioni mancanti, queste informazioni non sono state fornite.

la differenza quest'anno? Anche su invito del relatore, nel corso dei lavori in Commissione bilancio è stato richiesto al Governo di presentare la tabella mancante, che è stata fornita. fornita. Non so se questo sia un mezzo falso o una verità. So certamente che negli anni precedenti ci siamo trovati in presenza di quattro falsi veri! Tra l'altro, ho detto che è stata presentata per quattro anni su cinque la Nota di aggiornamento, poiché il quinto anno, cioè l'ultimo, ciò non è avvenuto. Mi permetto di avanzare qualche sospetto: forse la Nota di aggiornamento l'anno scorso non è stata presentata perché i conti erano troppo brutti ed era meglio evitare una discussione su questo aspetto. Credo che sarebbe meglio evitare troppa enfasi su questo aspetto, soprattutto perché vi sono colleghi che non è che nei quattro anni precedenti passassero per caso nel dibattito sulle leggi finanziarie: erano protagonisti di questo dibattito. Allora, forse sarebbe opportuno ricordarsi di quanto successo e collocare su un piano più serio,

È stato detto da molti colleghi che questa Nota di aggiornamento smentisce i luoghi comuni che la maggioranza aveva lanciato in questi mesi, e in particolare smentisce questi luoghi comuni, queste interpretazioni o questa enfasi sul versante sul versante dell'andamento dell'economia e su quello dell'andamento conti pubblici. Non è vero, dicono questi colleghi, che l'economia andava male, tant'è che la Nota di aggiornamento registra un suo miglioramento nel corso del 2006.

Presidente, lo stesso discorso vale per l'andamento dei conti. I colleghi sanno benissimo qual è stato il senso delle conclusioni della commissione Faini: il senso delle conclusioni della commissione Faini: sono i dati strutturali di andamento dei conti pubblici ad essere in difficoltà, più che i dati relativi agli andamenti congiunturali e dell'indebitamento.

nostro Paese. Lo stesso discorso vale per le scelte che sono state fatte e che restano nascoste. Ne cito soltanto una: c'è un'esigenza ordinaria e normale di trasferimento al settore delle ferrovie da parte del bilancio pubblico di 3 miliardi di euro. L'anno scorso la legge finanziaria ha ridotto 3 miliardi di euro a 300 milioni e abbiamo dovuto risolvere il problema con decreto-legge a luglio.

che le osservazioni che avevo svolto durante la mia relazione non abbiano trovato sufficiente smentita da parte dei colleghi della maggioranza. francamente non vorrei proseguire con considerazioni un po' tecniche ma soprattutto politiche che avevo fatto nel corso della mia relazione iniziale,

per l'aumento stesso della spesa, comporta, naturalmente, un considerevole aumento delle entrate attraverso l'imposizione di nuove tasse, sia dirette che provenienti da altre istituzioni della Repubblica, come le Regioni e, in particolare, i Comuni. Già in questa Nota di aggiornamento

Ieri, il ministro Padoa-Schioppa, nei lucidi che ha distribuito per la sua audizione, ha cifrato la manovra per 34,7 miliardi di euro.

il testo non ha ancora cominciato il suo *iter* emendativo parlamentare e dunque è lo stesso uscito dal Consiglio dei ministri. A parità di testo normativo, scopriamo però

Rimarrebbe sul piano della polemica politica. In verità, voglio chiedere al Governo di darci conto di come una manovra, a testi invariati, possa aumentare di 1,3 miliardi.

Se il nostro compito è di votare una Nota purchessia e delle tabelle purché siano, allora va bene, ma si comprende come la deliberazione parlamentare in tal modo viene svuotata di ogni contenuto e persino di ogni senso politico e normativo.

Nota di aggiornamento, chiedo formalmente che il Governo fornisca al Senato della Repubblica una spiegazione puntuale del perché, a testi invariati, l'entità della manovra sia mutata da 33,4 a 34,7 miliardi di euro.

e la Nota sul tendenziale, che è stata prodotta dalla mia persona a nome del Governo in quella sede. Intanto vorrei ricordare - com'è stato sottolineato nel corso dei diversi interventi, soprattutto da parte del senatore Morgando - che la Nota è pervenuta perché era doveroso che pervenisse,

ci sarebbe stato maggiore tempo a disposizione per quegli approfondimenti che sono stati richiamati come necessari da parte di molti senatori nel dibattito. quindi precisare che la Nota non è anonima, ma è autentica e, poiché risulterà prodotta nel resoconto della Commissione a mio nome, da me inoltrata, mi premeva chiarire questo punto. la discussione che svolgiamo sull'aggiornamento del DPEF, vorrei porre l'accento su alcuni punti che mi sembrano di particolare rilevanza. Il Governo

e che sono stati richiamati; anche ieri abbiamo ricevuto una particolare attestazione di interesse e di sostegno in Europa dal ministro Padoa-Schioppa in occasione della riunione che riguardava proprio la discussione sui conti. quindi di una manovra coerente con gli impegni assunti in sede europea e con la necessità di ridurre la spesa; per questo abbiamo posto l'attenzione su alcuni comparti importanti della spesa pubblica del nostro Paese. È vero che è in corso una discussione, che potrà, da qui all'approvazione della finanziaria, sicuramente produrre anche delle modifiche e degli aggiornamenti; ma il Governo è impegnato a produrre risultati rilevanti in questo senso. un intervento teso ad incidere fondamentalmente sulla riduzione del debito, che quindi libera risorse importanti per lo sviluppo e il rilancio del Paese. Come abbiamo detto più volte, è una manovra che vuole coniugare insieme risanamento, equità, crescita. Su questo argomento, vorrei anche aggiungere che siamo in una fase nella quale non ci possiamo permettere, data la situazione che abbiamo di fronte, di esercitare una politica dei due tempi, ma abbiamo bisogno di mettere insieme queste due azioni.

Ho sentito richiami particolarmente critici al lavoro della commissione Faini e al modo in cui il Governo nel suo insieme, ma anche il Ministro, ha

ma la constatazione di una situazione di particolare delicatezza alla quale occorre porre rimedio e che sarebbe sbagliato sottovalutare in questa sede per ragioni di interesse di parte. Una seconda questione riguarda la situazione relativa al debito pubblico, che nel 1992 era al 105,2 per cento e che attualmente, sia nella previsione del DPEF che nella ricognizione sui conti pubblici, supera

un impegno riformatore di questo Governo in materia di liberalizzazioni, di concorrenza, di sostegno allo sviluppo, di miglioramento del sistema delle infrastrutture del Paese. Voglio sottolineare, in proposito, che la

cantieri che figuravano finanziati ma non lo erano sostanzialmente. Quindi, c'è una barra, una direttrice, sulla quale siamo fortemente impegnati, che guarda fondamentalmente alla necessità di esercitare una politica di rigore insieme a quella di rilanciare un processo

decisamente negativi sia per quanto riguarda l'indebitamento sia per quanto riguarda la partita delle entrate. Questa previsione, però, è stata ampiamente affrontata nell'ambito del collegato fiscale, come è noto a tutti i senatori. Gli altri punti, invece, hanno un segno positivo e su di essi occorre concentrarsi con molta attenzione: mi sto riferendo al al tema della ripresa economica, e quindi ad un miglioramento delle previsioni di crescita del PIL del Paese, e soprattutto al rilevante importo del gettito, aumentato considerevolmente e sul quale evidentemente incidono diversi fattori

versamenti effettuati, si potrà fornire un dato sicuramente più aggiornato e più preciso di quanto non sia stato fatto in questa sede. In conclusione, riprendendo

un terreno di dialogo importante per riuscire a produrre, come risultato finale, una finanziaria che rispecchi fondamentalmente gli obiettivi dei quali abbiamo parlato e che trovi un livello di consenso e consapevolezza più forte nel Paese.

Signor Presidente, intervengo per ribadire ancora la nostra piena contrarietà, e quindi il voto contrario del nostro Gruppo, la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011; considerato (arrampicandovi sugli specchi per la quadratura di conti assolutamente privi di fondamento; basti pensare al buco di 17 miliardi, più del 50 per cento della manovra finanziaria, dovuto al rimborso dell'IVA, di cui non si parla in questa Nota di aggiornamento e di cui non si parla neanche nel rimborso della relativa copertura: sono 3,5 miliardi di mancata entrata e 3,5 miliardi di rimborso) si evince infatti soltanto un aumento di politiche basate prevalentemente sull'incremento del prelievo tributario a danno sia dei contribuenti, sia dell'impresa, con effettipenalizzati sull'intero sistema economico. Risulta da voi del tutto capovolto, come è tipico di taluni orientamenti comunisti, l'impianto del precedente Governo Berlusconi, che invece, come attestato proprio nella stessa Nota di aggiornamento, ha prodotto un miglioramento del PIL e un incremento complessivo delle entrate. Basti ricordare a tutti che agli inizi di quest'anno il Governo Berlusconi vi ha regalato un *surplus* di entrate di 20 miliardi di euro di cui non avete voluto assolutamente tener conto, preferendo un'operazione più facile: mettere le mani nelle tasche degli italiani. Ricordate che il DPEF e la stessa finanziaria che ci avete proposto, e che vi impediremo di approvare a tutti i costi, anche con manifestazioni di piazza,

sull'istigazione all'invidia sociale e sull'indicazione come colpevoli delle difficoltà economiche dei soggetti appartenenti al cosiddetto ceto medio e al campo delle imprese e del lavoro autonomo, che invece costituiscono i veri motori dell'economia.

interviene sul fatto che vi è un aumento incontrollabile - «non più controllabile» si dice - della spesa

del precedente Governo negli ultimi cinque anni. L'aumento della spesa corrente primaria si è verificato in modo particolare durante l'ultima legislatura, per circa 90 miliardi di euro. Mi sembra assolutamente contraddittorio che

prende a pretesto alcune valutazioni, che possono essere ascritte alla cosiddetta sinistra radicale, circa il fatto che la riduzione del cuneo fiscale è prevista solo per il sistema delle imprese e non è prevista, invece,

ai cosiddetti fondi chiusi gestiti dal sistema delle aziende e dalle organizzazioni sindacali. Se non interviene un chiarimento in proposito, il rischio molto reale è che non parta la previdenza integrativa nel nostro Paese e questo sarebbe un grave danno.

DPEF approvato è fondamentale per avere un quadro certo dell'andamento dei conti pubblici e le idee chiare relativamente ai provvedimenti da adottare. Le stime corrette saranno di giovamento all'intera manovra di bilancio, quest'anno particolarmente articolata e composita. Sì, perché accanto alla legge finanziaria sono previsti i Testi unici degli enti locali e sul federalismo fiscale, nonché tutta una serie di provvedimenti guida per la riorganizzazione della pubblica amministrazione, per lo sviluppo economico e per il completamento dell'opera di liberalizzazione. A partire dal cosiddetto decreto Bersani-Visco, questo Governo ha emanato, o sta per emanare, un complesso di norme che puntano a disegnare un Paese più moderno. Vediamo in prospettiva un'Italia dove si tende lentamente, ma con decisione, a decentrare sulle autonomie locali parti di spesa e d'entrata, mediante nuove forme d'imposizione fiscale o con partecipazione al gettito; il tutto mediante un patto di responsabilizzazione che lega autonomie e Stato centrale, a beneficio del cittadino. Ecco perché dobbiamo registrare con favore i dati contenuti nella nota relativa al maggior gettito delle entrate tributarie, circa 6 miliardi, in quanto derivante da un allargamento della base imponibile, ovvero dall'aumento dei contribuenti che pagano le tasse. La progressione strutturale di buona parte di questo gettito - 5 dei 6 miliardi di maggior gettito complessivo - è certamente un dato positivo che gioverà significativamente significativamente sui provvedimenti che compongono complessivamente la manovra di bilancio. Sul punto dei rapporti con le istituzioni europee, il dato negativo, derivante dalla sentenza sulla detraibilità dell'IVA, viene neutralizzato dal giudizio positivo sull'IRAP, anche se è chiaro che le due imposte impattano sul bilancio con cifre differenti. In termini di saldi, tuttavia, si registra un minor gettito di circa 3,7 miliardi di euro per l'IVA sulle auto nel 2006 e maggiori oneri per il periodo pregresso 2003-2005 per 13.400 milioni Questo dato tutto negativo inciderà sui conti dei prossimi esercizi finanziari, si registra però l'amarezza per il fatto che al netto di debiti pregressi, con la sentenza sull'IVA, già dal 2006 avremmo potuto ridurre l'indebitamento ad una cifra vicina al 3 per cento. Allo stato dei fatti, viceversa, l'indebitamento sarà pari al 4,8 per quest'anno, con l'obiettivo di scendere al di sotto del 3 per cento nel 2007, per arrivare allo 0,1 nel 2011. Resta fermo l'intento di ridurre il debito pubblico al 97,8 per cento rispetto al PIL del 2011. In ogni caso, il dato politico che emerge è quello di una manovra di bilancio che, sin dai dati di questa Nota, si presenta come complessivamente apprezzabile per lo sforzo che mette in atto. Per quanto ci riguarda, sin d'ora rileviamo che il riequilibrio finanziario non può penalizzare le famiglie del ceto medio, peraltro coinvolte e poco tutelate dalla manovra. Perciò su questo chiederemo modifiche tangibili e penso che gli alleati del centro-sinistra comprenderanno la necessità di tali aggiustamenti

e firma mia e del collega Forte, a nome dell'UDC. Tale orientamento negativo verso la Nota di aggiornamento è motivato da due ragioni: la prima, di natura tecnica, perché la Nota la funzione che la normativa contabile le attribuisce, vale a dire di aggiornare i dati relativi al quadro macroeconomico e di finanza pubblica in relazione all'evoluzione degli andamenti e non assolve a tale compito. La Nota, invece, corregge di fatto in modo significativo gli obiettivi stabiliti dal DPEF di luglio in quanto macroscopicamente errati, come già detto in discussione generale, perché basati su una *due diligence* fortemente politicizzata. La seconda ragione è politica: la Nota risponde ad un'esigenza politica, imposta dalla sinistra radicale, di definire una manovra correttiva tutta improntata sulla leva fiscale e priva di quelle riforme strutturali preannunciate nel DPEF di luglio.

«per la parte di contenimento del disavanzo tendenziale essa» - la manovra - «interesserà necessariamente anche il lato della spesa e consisterà di provvedimenti riformatori di carattere strutturale che interverranno anche sui quattro grandi comparti della spesa pubblica (pubblico impiego, previdenza, sanità, finanza territoriale)». Niente di tutto questo figura nella finanziaria 2007 e nella Nota in discussione. Avevate scritto che il cuneo fiscale avrebbe agito anche sul miglioramento della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Invece niente, nemmeno un rigo. Niente per l'occupazione delle donne. Ai giovani assunti con la legge Biagi avete aumentato la quota contributiva, senza rimuovere la sofferenza delle «pause» di lavoro, sulle quali avete costruito tutta la vostra campagna elettorale. Niente potenziamento dei servizi per l'infanzia. Niente *fiscal* *drag*. Niente aumenti degli assegni familiari per i figli dei lavoratori autonomi e dei disoccupati. premessa della risoluzione di luglio, avevate scritto: «sostenere i redditi di quanti vivono rapporti di lavoro discontinui e/o con basse retribuzioni»; invece, avete fatto l'opposto; niente per gli incapienti, cioè per coloro che non possono beneficiare degli sgravi fiscali perché non soggetti a tassazione. Tagli alla scuola. Tagli alla sanità. Tagli alla pubblica sicurezza. Tagli alla giustizia. Tagli ai servizi sociali. Avete aumentato le spese militari, voi marciatori della pace. Ma che razza di sinistra è questa che governa l'Italia? Avete dato con la mano destra qualche euro in più ai redditi sotto i 20.000 euro, ma ve li siete ripresi qualche riga dopo nella finanziaria con la tassa di scopo, con l'aumento dell'ICI e delle rivalutazioni catastali, della compartecipazione IRPEF per gli enti locali, con l'aumento dell'accisa sulla benzina e del bollo per chi non ha potuto rinnovare l'auto perché a basso reddito. *E* del dispositivo della vostra risoluzione del DPEF di luglio, che era necessario «rafforzare gli strumenti per la conciliazione tra vita lavorativa e vita personale e familiare», ossia sostenere la donna e la madre che lavora. Ditemi quale rigo, quale norma della finanziaria 2007 e dei provvedimenti collegati parlano di questo impegno. Avevate preso impegni nella vostra risoluzione a favore del reddito minimo di inserimento; aiutateci a cercarlo

e invece avete cancellato la norma del cinque per mille della finanziaria dell'anno scorso. Abbiamo presentato una risoluzione incentrata sulla famiglia:

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor membro del Governo, il voto della Lega Nord è un voto contrario e convinto alla proposta di risoluzione

che in questi giorni sta trovando riscontro molto forte in larga parte del Paese, nel ceto produttivo, ma anche nel ceto medio-basso. Dal punto di vista tecnico avevamo già ricordato che il Governo aveva dichiarato che i 33,4 miliardi sarebbero stati ottenuti per un terzo con aumento di tasse e per due terzi con tagli alla spesa e destinati, rispettivamente, per un terzo al taglio del *deficit* pubblico per due terzi allo sviluppo e all'equità**.** Abbiamo già sottolineato nella relazione, facendo eco anche ai colleghi, che i 5 miliardi di TFR trasferiti all'INPS non sono tagli di spesa, ma sono spostamento di patrimonio dai lavoratori allo Stato. Questo è un dato politico importante. Siamo passati, ripeto agli amici della sinistra (mi riferisco in particolare ad alcuni settori sicuramente oggi rappresentati), dall'esproprio proletario all'esproprio ai proletari.

anche con l'intervento per quanto riguarda l'IRPEF. Avevate fatto credere alla base elettorale che solo i ricchi avrebbero pianto e invece la soglia dei ricchi si abbassa sempre di più e

che ha un coniuge e figli a carico, scontando l'incremento delle deduzioni, subirà un aumento di tassazione. Per non parlare del partito delle tasse che si è formato, molto unito, e che non ci potrà mai vedere in qualche modo uniti perché «basta Roma, basta tasse» vale ancora oggi per il Nord e anche per questa parte dell'opposizione che vuole segnalare come gli aumenti surrettizi per l'IRPEF e per l'ICI andranno a penalizzare pesantemente una parte dei lavoratori e influiranno sugli investimenti in modo chiaro. Anche sulla destinazione delle risorse, sulla riduzione

l'aumento delle tasse, mentre per la crescita registriamo una minore crescita del PIL. Crediamo sia importante verificare anche a livello europeo; noi auspichiamo un controllo europeo rigoroso. Ricordo che nella scorsa finanziaria eravamo presidiati dall'Unione Europea nel Ministero e non potevamo pensare ad alcun emendamento

quello che sarà il *deficit* dell'IVA e scaricate quello che è in conto capitale, la crescita nei prossimi quattro-cinque anni, voi già oggi mettete un'ipoteca e fate il

porteranno un risultato elettorale, quanto meno mediatico, ma siamo coscienti e siamo convinti che gran parte del ceto medio, quello che si è espresso a favore magari anche della formazione della Margherita,

che, tra l'altro, affronta l'annoso problema della titolarità della convocazione delle assemblee in orario di lavoro da parte delle organizzazioni sindacali che presentano liste per le elezioni delle RSU. L'urgenza della risposta è data dall'imminente rinnovo delle RSU nella scuola, in vista del quale alcune sigle, anche storiche, del mondo sindacale e scolastico sono tuttora escluse da tale diritto. Alcuni esponenti, in particolare del COBAS della scuola, da dieci giorni sono in sciopero della fame davanti alla sede del Ministero della pubblica istruzione per ottenere un minimo di equità di trattamento. Alcune trattative erano state avviate